sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. Senatori, il 6 aprile 2009, alle ore 3,32 della notte, una terribile scossa di terremoto sconvolse la città dell'Aquila, l'Abruzzo e tutto il Centro Italia. Sotto le macerie rimasero bambini, ragazze e ragazzi, intere famiglie, anziani, soccorritori. Il bilancio finale fu drammatico: persero la vita oltre 300 persone, con più di 1.500 feriti e decine di migliaia di sfollati. Tra le vittime permettetemi di ricordare Giovanna Berardini, giovane mamma, che il giorno dopo avrebbe dovuto partorire la sua seconda figlia, Giorgia. Il terremoto portò, invece, via l'intera famiglia, compreso il figlioletto Francesco di due anni. E poi case, scuole, chiese, edifici pubblici; il centro storico e le zone più colpite furono distrutte in pochi secondi, cancellando per sempre storie, ricordi, affetti, volti. La macchina dei soccorsi restituì al Paese quella dignità e quell'orgoglio che la tragedia aveva messo a dura prova. Da tutta l'Italia ci si mobilitò per aiutare, sostenere, confortare quei connazionali che avevano perso tutto; una gara di solidarietà, alla quale parteciparono anche Stati esteri, fondazioni, organizzazioni internazionali. A distanza di dieci anni abbiamo il dovere morale di ricordare e abbiamo l'obbligo di ispirare ogni giorno le politiche pubbliche ai princìpi di sicurezza del territorio e dell'ambiente. In ricordo delle vittime, vi invito ad un minuto di raccoglimento.

finestra") sull'immobile da destinare a nuova sede della questura di Pesaro. gli uffici della questura di Pesaro e Urbino sono ubicati in differenti immobili, detenuti in regime di occupazione extracontrattuale, con sede centrale in via Giordano Bruno e una seconda sede, ubicata in via Flacco, adibita a sede degli uffici immigrazione e personale. Con riferimento a questo secondo immobile, di proprietà di una società interamente partecipata dalla Provincia di Pesaro e Urbino, è stata anche attivata una procedura di sfratto per finita locazione con rilascio previsto, dopo due intervenute proroghe, alla fine del 2019. Al fine di individuare soluzioni alternative idonee a sistemare gli uffici attualmente dislocati nell'immobile di via Giordano Bruno, la prefettura, in stretto raccordo con la questura e l'Agenzia del demanio, ha avviato, fin dal 2015, le procedure per rendere possibile il recupero, con oneri a carico dell'Agenzia del demanio, di un immobile demaniale, adiacente alla sede della prefettura, un tempo sede dell'Intendenza di finanza e del Comando provinciale della Guardia di finanza, da anni inutilizzato. Nel nuovo stabile saranno allocati parte degli uffici attualmente situati nella sede principale di Via Giordano Bruno e sarà ricavata un'area interna per lo stazionamento delle autovetture di servizio. Gli uffici di Via Flacco, invece, saranno trasferiti nell'attuale edificio principale della questura, che si trova nella medesima piazza in posizione frontale ed a poche decine di metri dal nuovo edificio. Tale ipotesi di risistemazione logistica si è concretizzata in un protocollo d'intesa, sottoscritto in data 17 giugno 2016, tra il Ministero dell'interno, l'Agenzia del demanio ed il Comune di Pesaro. In particolare, la citata Agenzia si è impegnata a progettare ed attuare l'intervento di adeguamento e ristrutturazione edilizia, per una spesa complessiva di 6,2 milioni di euro, ed ha elaborato un progetto definitivo degli interventi, che include anche opere di riduzione del rischio sismico. Ai fini della stesura della progettazione esecutiva è stato elaborato un apposito programma, approvato dalla Soprintendenza ai beni artistici e culturali, per il posizionamento di alcuni *container*, strumentali alla temporanea collocazione dei negozi sulla piazza antistante l'edificio nel periodo necessario alla esecuzione dei lavori. Proprio con riferimento alla presenza degli esercizi commerciali posti al piano terra dello stabile va evidenziato che la situazione era nota all'atto della stipula del protocollo d'intesa nel 2016 a tutti gli uffici locali, interregionali e centrali interessati, che hanno valutato positivamente l'intervento sotto il profilo della funzionalità, ritenuta in linea con le regole tecniche e amministrative dettate per gli interventi del tipo innanzi prospettato. Si evidenzia, inoltre, che i suddetti esercizi commerciali non sono comunque situati a ridosso degli ingressi principali, né della prefettura né dello stabile individuato per il trasferimento degli uffici della questura. L'attuazione dell'iniziativa in parola viene, peraltro, costantemente monitorata da un apposito gruppo di lavoro composto, come indicato dal citato protocollo d'intesa, da rappresentanti delle parti sottoscrittrici, nonché da un referente locale del Dipartimento della pubblica sicurezza territorialmente competente, che garantirà il necessario supporto tecnico all'Agenzia del demanio affinché il relativo progetto di adeguamento sia conforme alle esigenze degli uffici di Polizia. L'iniziativa in questione, il cui termine presumibile di ultimazione dei lavori è previsto per la fine del 2021 o l'inizio del 2022, si presenta economicamente vantaggiosa per l'amministrazione, in quanto, essendo l'immobile demaniale, non dovranno essere corrisposti canoni e le opere di adeguamento alle esigenze di Polizia saranno realizzate e finanziate dall'Agenzia del demanio. Si fa presente, da ultimo, che non risultano finora pervenute proposte in merito alla realizzazione di una nuova struttura sull'area edificabile di proprietà del Comune, adiacente il parco Miralfiore, soluzione che comunque non sarebbe economicamente più vantaggiosa, dovendo il Ministero dell'interno in tale ipotesi corrispondere un canone di locazione per l'utilizzo dell'immobile che il Comune di Pesaro andrebbe a realizzare. La prefettura di Pesaro e Urbino ha peraltro fatto sapere che in una delle ultime riunioni del Consiglio comunale di Pesaro è stato respinto a maggioranza un ordine dei giorno presentato da un consigliere di minoranza con il quale si impegnava l'amministrazione comunale a trovare altre soluzioni per l'allocazione della questura.

un'interrogazione che nasce dal doveroso rapporto tra parlamentari e territorio che li ha espressi. Mi sono fatto carico dei dubbi manifestati da un sindacato di Polizia, dubbi che hanno animato un dibattito sui giornali cittadini, a seguito del quale diversi cittadini mi hanno scritto aderendo a questi dubbi e sollecitandomi a prendere una posizione. Prendo atto della cronologica ricostruzione dei fatti svolta dal sottosegretario Molteni, che mi pare non aggiunga valutazioni di merito alla scelta fatta dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci. scelta è, a mio avviso, discutibile per tante ragioni: in primo luogo per questioni di sicurezza. Ne ha fatto cenno il Sottosegretario: i negozi che si trovano al piano strada espongono al rischio e favoriscono l'intenzione di eventuali malintenzionati che volessero fare un attentato alla questura. La nuova questura si troverebbe poi collocata nel pieno del centro storico cittadino, zona a traffico limitato, a ridosso di Piazza del Popolo, frequentatissima dai pesaresi, i quali ritengono giustamente un loro diritto passeggiare in serenità. che mal si concilierebbe con il viavai di volanti di Polizia che fanno il loro mestiere, ma metterebbero anche a rischio la sicurezza dei cittadini che lì passeggiano. La struttura individuata, inoltre, proprio per la sua morfologia, non pare adeguata alla funzione che andrebbe a ricoprire. Non si libererebbe automaticamente la vecchia questura e quindi ci sarebbe una coabitazione di uffici in edifici diversi, cosa che immagino non possa favorire la funzionalità del lavoro di chi all'interno della nuova questura. Non ci sono poi parcheggi, e questo penalizza i dipendenti della questura, così come i cittadini chiamati a frequentarla. Meglio sarebbe stato, a mio avviso, utilizzare il terreno di proprietà del Comune cui lei ha fatto riferimento - 20.000 metri quadri edificabili - per costruire una nuova questura con tutti i crismi e, dopo un accordo con il demanio, restituire alla città l'edificio dell'ex Intendenza di finanza perché, come sappiamo, Pesaro è una città ricca di fermento culturale e associativo ma povera di luoghi dove tale fermento possa realizzarsi, svolgersi, aprirsi effettivamente alla cittadinanza. Quindi, dal mio punto di vista, meglio sarebbe stato, per la collocazione di quell'edificio (l'ex Intendenza di finanza) per la sua struttura, aprirlo e restituirlo effettivamente alla cittadinanza piuttosto che trasformarlo in una questura, o meglio in una mezza questura, dal momento che una parte della vecchia questura resterebbe in funzione. Comunque, *ubi maior*, prendo atto della posizione del Governo e dell'amministrazione comunale di Pesaro e speriamo che si riveli la scelta giusta.

il senatore Quarto chiede notizie relative all'istituzione di un Archivio di Stato nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Vorrei premettere che, come correttamente ricordato dal senatore interrogante, il decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963, che detta norme relative all'ordinamento del personale degli archivi di Stato, prevedeva un Archivio di Stato in ogni provincia, con sede nel capoluogo. La competente Direzione generale del Ministero per i beni e le attività culturali, già nel marzo del 2008, aveva espresso la propria disponibilità ad attivarne uno nella provincia in parola, purché gli enti locali si fossero fatti carico dei problemi connessi all'adeguamento strutturale e funzionale delle sedi, tenuto conto delle difficoltà di bilancio evidenziate anche dagli altri uffici del Ministero presenti sul territorio. La stessa Direzione archivi, su impulso del segretario generale che si era fatto interprete della richiesta avanzata in tal senso dal commissario governativo per la Provincia di Barletta-Andria-Trani, provvide a quantificare gli oneri necessari per l'attivazione e il successivo funzionamento dell'Archivio di Stato di Trani, addivenendo alla conclusione che non sarebbe stato possibile farvi fronte con le risorse ordinarie. Si conviene con il senatore interrogante circa il fatto che la presenza di personale d'archivio già addetto al servizio presso le sezioni distaccate non comporta, per tali voci di spesa, oneri aggiuntivi e tuttavia la funzionalità di una serie di archivi esige una più complessa organizzazione anche strutturale. Nell'ampio confronto che ha riguardato la valutazione delle ragioni culturali dell'iniziativa, ma anche le sue implicazioni finanziarie, organizzative e logistiche, si è ritenuto di mantenere per ora l'assetto esistente, con gli uffici di Barletta e Trani come sezioni dell'Archivio di Stato di Bari. Nel 2016 sono stati assegnati, per l'adeguamento strutturale e funzionale della ex caserma Stennio di Barletta 974.500 euro complessivi di cui 706.500 euro imputabili alla programmazione ordinaria dei lavori pubblici e 268.000 euro stanziati con legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tale somma non è tuttavia sufficiente per ultimare i lavori necessari. Vorrei infatti rammentare che già nel 2008 l'ufficio tecnico della competente Direzione generale archivi aveva stimato l'importo necessario all'adeguamento strutturale in 2,5-3 milioni di euro. È stato quindi previsto di realizzare in via prioritaria gli interventi comunque necessari per avviare la procedura di messa in esercizio dell'attività nel rispetto

le città di Barletta e di Trani circa l'ubicazione della sede principale dell'istituendo Archivio di Stato. Vorrei tuttavia rassicurare il senatore interrogante che il Ministero per i beni e le attività culturali, che, tra le altre, svolge le funzioni statali relative alla tutela del patrimonio archivistico italiano e ne promuove la conservazione, la conoscenza e lo studio, è ben consapevole dell'importanza degli Archivi, sono un bene prezioso e delicato dove lavorano professionisti che conservano il passato e organizzano il presente, permettendo a tutti di usufruire di inestimabili documenti che essi stessi salvaguardano per il futuro, e persevera nella ricerca di ogni possibile soluzione per realizzare quanto richiesto; una soluzione che contemperi e soddisfi il piano culturale e quello finanziario nel quadro di un piano di riorganizzazione del Ministero. Signor Presidente, esprimo la mia soddisfazione per questa circostanziata e completa risposta del Governo. Finalmente, dopo quindici anni dalla nascita della Provincia di Barletta-Andria-Trani, si prende seriamente in considerazione l'istituzione della sede provinciale dell'Archivio di Stato, così come prevede la legge dello Stato. Raccogliere, conservare e sorvegliare il patrimonio archivistico e documentario di proprietà statale e renderlo fruibile ai cittadini: è questo l'importante compito degli Archivi di Stato. Preziosa risulta l'assistenza ai ricercatori in sala studio e le ricerche per corrispondenza, l'acquisizione della documentazione storica degli uffici statali, l'attività promozionale e didattica, le iniziative di ricerca scientifica e di valorizzazione dei documenti, anche in collaborazione con altri istituti culturali. Tutto ciò è sicuramente più efficiente se nel territorio esiste una sede provinciale. Per troppo tempo i Governi precedenti hanno ignorato questa legittima istanza che - sia chiaro - non comporterebbe oneri aggiuntivi. Sono infatti già operative sul territorio, come sezioni dell'Archivio di Stato di Bari, le sedi di Barletta e Trani, dotate nel complesso di circa 100.000 documenti di interesse archivistico, atti di carattere amministrativo, finanziario, giudiziario e militare, in alcuni casi risalenti al XVI secolo. Sul piano delle risorse umane poi queste due sezioni hanno già una qualificata e completa dotazione tra funzionari archivisti e addetti ai servizi e possono usufruire di due splendidi edifici, ricordati anche dal Sottosegretario: l'*ex* caserma Stennio di Barletta, un tempo convento dei Celestini, le cui prime notizie riguardanti la chiesa con l'annesso monastero e ospedale risalgono al 1185, e lo storico palazzo Valenzano di Trani, risalente al 1762, già sede dell'archivio notarile distrettuale. Ho fatto presente nell'interrogazione che la provincia di Fermo, nata anch'essa nel 2004, ha ottenuto la trasformazione da sezione di Archivio di Stato in Archivio di Stato di Fermo già nel 2007. Credo sia giunto il momento di procedere anche nella sesta provincia pugliese. Il Ministero per i beni e le attività culturali potrà quindi indicare come sede Barletta o Trani. Approfitto dell'occasione per sollecitare tutti gli enti coinvolti ad accelerare le procedure per completare i lavori di adeguamento e di messa in sicurezza delle strutture che ospitano o ospiteranno a breve i documenti archivistici. Il Governo, dal canto suo, deve impegnarsi ad agire tempestivamente appena il territorio sarà pronto con una sede ad accogliere l'Archivio di Stato. Vorrei salutare i rappresentanti delle Consulte degli studenti del Friuli-Venezia Giulia.

l'ufficio della motorizzazione civile (UMC) di Prato, nel dicembre 2012, è stato chiuso anche a seguito delle misure contenute nel decreto-legge n. 95 del 2012, con conseguente accorpamento all'UMC di Firenze. I pensionamenti, il blocco del *turnover* e la rotazione di personale hanno determinato criticità nell'erogazione del servizio. Con riferimento al periodo di validità del foglio rosa, la circolare ministeriale del 2 marzo 2016 ha fornito disposizioni in relazione alla possibilità di proroga. Evidenzio, inoltre, che un'apposita commissione ispettiva del MIT, nominata nel 2018 per verificare le effettive situazioni di criticità lamentate dalle autoscuole, ha riscontrato che la cosiddetta vita media del foglio rosa di Firenze è di circa cento giorni, cioè in linea con la media nazionale. Al riguardo, informo che a febbraio 2018 è stato assunto un funzionario ingegnere nell'ufficio di Firenze, mentre per le future assunzioni di personale a tempo indeterminato presso il MIT, una parte considerevole delle stesse sarà effettuata tramite apposito concorso a 148 posti di funzionario ingegnere architetto - di cui cinque per la Motorizzazione di Firenze e le relative sezioni - le cui prove scritte si sono già svolte; al riguardo, si è già richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze la possibilità di prevedere, con il primo strumento normativo utile, un incremento dei posti già messi a concorso. Aggiungo anche che, sempre per la carenza del personale della Motorizzazione, in manovra è stato inserito un fondo da 16 milioni di euro, ovviamente spalmato su vari anni, per ulteriori cinquanta assunzioni per venire incontro a questa carenza evidente che abbiamo ereditato. Proprio per far fronte alle richieste dell'utenza si sta intervenendo attraverso miglioramenti organizzativi. L'attività operativa viene anche soddisfatta grazie ad una maggiore presenza, in regime di straordinario, da parte del personale dell'ufficio. È comunque allo studio, tra le misure da inserire nelle proposte di legge di modifica al codice della strada, quella della proroga del foglio rosa, quando al candidato non è dato di sostenere le due prove di esame di guida in costanza di validità della certificazione, misura che, quindi, permetterà di abbattere i costi del rinnovo del foglio rosa. Alla luce di quanto esposto, rassicuro che la competente Direzione generale territoriale svolge e continuerà a svolgere la propria attività di monitoraggio sulle criticità lamentate e cercherà di assumere tutti i necessari provvedimenti. Infine, informo che in ogni sede periferica sono in fase di attivazione corsi di abilitazione per l'espletamento

Anche considerato il fatto che l'interrogazione risale a molti mesi fa, ho potuto fare nuove verifiche con gli operatori e con i cittadini che avevano sollevato la questione e denunciato l'esistenza di un problema grave. Da queste verifiche è emerso che il quadro che attualmente abbiamo per quanto riguarda la Motorizzazione di Firenze e Prato è molto meno roseo di quello che ci viene descritto e che le prospettive non sono affatto favorevoli come quelle che lei ci ha prospettato. Sappiamo bene che c'è stata una svolta in questa vicenda che si è verificata nel mese di aprile del 2018, quando è stato rimesso in discussione un accordo precedente; ciò ha determinato una grave ricaduta sul servizio. Sappiamo che per molto tempo si è andati avanti con un grande sacrificio dei cittadini e degli operatori professionali, che hanno cercato di supplire con la loro buona volontà agli effetti gravi delle carenze di organico. Sappiamo anche che i rimedi strutturali che occorrono per poter avviare veramente a soluzione questo problema sono di dimensioni assai più ampie rispetto a quelle dei rimedi che lei ha accennato. Comunque, apprezzo il tentativo di mettere in campo una soluzione. Registro il suo ottimismo sull'effetto che avranno le iniziative in corso. Le ricordo soltanto che le assunzioni programmate sono, a mio parere, davvero insufficienti a mutare la situazione nella Motorizzazione civile di Firenze e Prato. L'esistenza di disagi così gravi come quelli che nella mia interrogazione sono riportati non è affatto attenuata dal constatare che la durata del foglio rosa in questa circoscrizione è la stessa che esiste, in media, nelle altre circoscrizioni, perché in questi casi mal comune mezzo gaudio non è un principio che vale. Mal comune è mal comune e non c'è altro da dire. Le dico anche che sarebbe bene che il Governo, come già avvenuto per ciò che concerne gli organici delle forze di polizia, desse un'informazione corretta sull'effetto, come saldo netto, dei concorsi che sono in programma. Infatti se, come da molte voci allarmate mi viene fatto sapere, ci sarà - all'interno di queste strutture - un ricorso massiccio alle nuove disposizioni sull'anticipo pensionistico, corriamo il rischio che l'immissione in ruolo di unità in più che lei ha ricordato alla fine porti a un saldo netto di personale in calo per l'effetto di un'altra misura che ha operato lo stesso Governo del quale lei è esponente e al quale appartiene. Anche in questo caso bisogna che la mano destra sappia quello che fa la mano sinistra, altrimenti non si riesce

il Governo italiano segue con grande attenzione la vicenda dell'avvocatessa iraniana Nasrin Sotoudeh e del marito Reza Khandan, sia direttamente che in coordinamento con i *partner* europei. Sul piano bilaterale, il ministro degli affari esteri Moavero Milanesi ha effettuato un passo formale con il proprio omologo iraniano, cui è stato anche confermato l'elevato interesse dell'opinione pubblica e delle associazioni professionali forensi italiane al caso, e con l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione europea Mogherini, affinché alla vicenda dell'avvocatessa Nasrin Sotoudeh sia dedicata la massima attenzione. Ancor prima della recente condanna, abbiamo preso parte attiva alle principali occasioni di discussione della situazione dei diritti umani in Iran nei competenti *fora* multilaterali. Da ultimo, nell'ambito dei lavori del Consiglio per i diritti umani dell'ONU a Ginevra, di cui l'Italia è parte, in occasione del dialogo interattivo con il relatore speciale ONU sulla situazione dei diritti umani in Iran (11 marzo 2019), l'Unione europea ha attirato l'attenzione, tra l'altro, sul forte impegno per la protezione e promozione della libertà di opinione, espressione, associazione e riunione. Allo stesso tempo, ha espresso forte preoccupazione per i continui arresti e detenzioni di persone che esercitano questi diritti, inclusi giornalisti, attivisti, avvocati e difensori dei diritti umani, così come di avvocati che difendono queste persone, sollecitando il Governo iraniano a rivedere le proprie politiche, azioni e leggi per assicurare la protezione di tali diritti. L'Unione europea ha inoltre sollecitato il Governo iraniano ad adottare ulteriori misure per garantire il pieno godimento dei diritti umani di donne e ragazze. A seguito dell'annuncio della recente condanna di Nasrin Sotoudeh, alla nostra ambasciata a Teheran è stato chiesto di coordinarsi con le altre rappresentanze dell'Unione europea accreditate nel Paese anche per chiarire i termini della pena inflitta, sui quali vi è divergenza tra quanto dichiarano ufficialmente le autorità iraniane (sette anni) e quanto dichiarato dalla famiglia (38 anni e 148 frustate). Si tratta di un accertamento non semplice, alla luce di alcune rigidità che sussistono nel contesto iraniano. Continueremo a sostenere le iniziative pianificate dall'Unione europea, che - ricordo - si è immediatamente attivata con una dichiarazione (il 12 marzo) nella quale si esprime preoccupazione per la condanna dell'avvocatessa. Allo stesso tempo, si richiama l'attenzione delle autorità iraniane sulle violazioni al diritto a un giusto processo subite dall'avvocatessa e sul fatto che il diritto di protestare ed esprimere pacificamente le proprie idee è sancito dal Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, di cui anche l'Iran è parte, e si chiede con fermezza l'immediata revisione della sentenza relativa all'avvocatessa e di quella del marito, oltre al rispetto del loro diritto di appellarsi contro le sentenze. Monitoreremo gli sviluppi futuri del caso, evocandolo con preoccupazione nei prossimi contatti bilaterali con Teheran e assicurando che esso sia approfondito dai competenti organismi multilaterali. Il binario multilaterale appare infatti la cornice più adeguata nella quale poter iscrivere, in coordinamento con i *partner* dell'Unione europea, azioni di pressione sulle autorità iraniane sia relative al caso specifico sia - più in generale - per stimolare risposte costruttive in tema di rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, inclusi quelli delle donne, da parte del Governo iraniano.

il re mettendosi alla guida della loro automobile; c'è una fortissima richiesta di scolarizzazione, attraverso la quale molte donne cercano di ottenere diritti

Sappiamo che a lei è stato applicato il massimo della pena su sette reati, che sono tutti discutibili perché bisognerebbe capire se realmente la condotta cioè, il fatto oggetto del reato, sia stata commessa da Nasrin. Soprattutto, è stato utilizzato un articolo del codice penale che, prevedendo il cumulo delle pene, prescrive l'applicazione di una norma aggravante che aumenta ulteriormente la pena. È ridicolo sostenere che non si possa accertare realmente il contenuto della sentenza: il Governo dice che è stata condannata a sette anni, ma sappiamo che è stata condannata a La certezza della pena dovrebbe essere uno dei fondamenti di uno stato di diritto. Sappiamo che, di fatto, abbiamo a che fare con un Paese dove lo stato di diritto è messo continuamente in discussione. tutte le iniziative di cooperazione internazionale che vengono comunque sostenute rispetto a quel Paese devono, possono, saranno - me lo chiedo e lo chiedo al Governo

chiedendo al Governo in cambio che vengano rispettati questi punti. Rispetto alla sua risposta, signor Sottosegretario, della quale la ringrazio, vedo delle lacune e, soprattutto, una mancanza di iniziativa politica molto forte. Abbiamo Ministri visibili che continuamente, anche con frasi fatte e *slogan*, lanciano sfide europee e internazionali, ma non vedo la stessa veemenza, la stessa presenza e lo stesso uso di un linguaggio forte e chiaro quando si tratta di difendere una donna, i diritti umani di una donna e, soprattutto, un'ingiustizia che ormai è sotto gli occhi del mondo.

c'è la sentenza del giudice (per inciso, il giudice che ha adottato questa sentenza è stato promosso all'ONU per occuparsi delle questioni femminili!).

Una comunità è fatta di leggi, reddito e ambizioni, ma anche di memoria collettiva. La memoria collettiva consente resistenza e resilienza quando si presentano difficoltà, situazioni di dolore e anche incertezze nella condotta, perché è più grande la difficoltà da gestire. L'Aquila ha conosciuto un terremoto di proporzioni anche scientificamente mai avvertite in quella parte di territorio del centro dell'Italia, se non si torna indietro al 1703. Come lei ha detto, signor Presidente, vite umane sono state colpite da un terremoto contro L'Aquila e non della città dell'Aquila. Il terremoto lascerà il ricordo del dolore per decenni, esattamente come accaduto nel 1703, quando ci fu un'identica scossa che distrusse il suolo e il sottosuolo, ma anche il cielo, a livello delle ambizioni. A che serve ricordare, in un momento come questo? Serve a prendere le misure circa le cose fatte, ma - soprattutto - a stabilire un livello collettivo di maturità, anche all'interno dell'ordinamento. Noi dobbiamo produrre una norma quadro riguardante i disastri, che non determini ogni volta il tiro alla fune per avere risorse

All'Aquila stiamo rivedendo le mura; stanno tornando le mura, anche più belle di quelle che c'erano in passato. Il problema è che quelle mura non raccontano vita, né ambizione e c'è bisogno di far sì che tornino anche la vitalità economica, culturale, solidale e la fiducia. Come avrebbe detto Pannella, che è stato e rimane un grande abruzzese, c'è bisogno di pertinacia - la tenacia pertinente, la pertinenza nella tenacia - di tutti coloro i quali hanno dovere. Ricostruire

ma in anticipo, prima che i disastri accadano. In quest'Aula un grande senatore, Gianfranco Miglio, ci ha spiegato che lo Stato si fa riconoscere se sa reagire ai disastri. Per queste ragioni ricordare torna utile, perché è una premessa per la nostra pertinacia. Grazie, signor Presidente. Grazie, Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, il 6 aprile ricorre il decennale di un evento tragico, tanto tragico e tanto lontano nel tempo eppure ancora così attuale. Nella notte tra il 5 e 6 aprile di dieci anni fa, alle ore 3,32, un boato avvolse la città dell'Aquila, un boato che riecheggia ancora in alcune di quelle strade che ancora oggi appaiono così come il terremoto le ha lasciate e ridotte: un cumulo di macerie. Bastarono pochi secondi, pochi interminabili secondi per stravolgere la vita di tante famiglie e far crollare i loro sogni, le loro certezze e le loro vite. 80.000 gli sfollati, 1.600 i feriti e 309 le vittime: questo è il rapporto del tragico evento. Sono passati dieci anni e a all'Aquila ci sono ancora 4.200 nuclei familiari in attesa di rientrare nelle proprie case; infatti, la ricostruzione risulta ancora distante dalla sua frase conclusiva, mancando all'appello ancora il 25 per cento di abitazioni nel centro, il 45 in periferia e ben il 78 per cento nelle frazioni. Dieci anni di attesa sono troppi ed è nostro compito oggi cercare di alleviare il dolore di tutti i cittadini aquilani e di tutti quelli che vivono la medesima situazione. Siamo tenuti a farli tornare a vivere nei propri quartieri, con le proprie abitudini e con le proprie comunità, a ridare loro una vita normale. Le stesse immagini di quel tragico 6 aprile si sono ripetute poi nel maggio del 2012 in Emilia-Romagna e, ancora, nel 2016 ad Amatrice. Per una Nazione che si rispetti frasi del tipo: «Si poteva evitare» oppure: «Si doveva intervenire prima» hanno il suono di una sconfitta, di un'incapacità dello Stato a fare lo Stato. Ogni vittima del terremoto è una parte di Stato che muore. È vero, l'Italia è una Nazione che ha sempre tremato e continuerà a farlo e, purtroppo, i terremoti non sono prevedibili, ma è altrettanto vero che abbiamo oggi le conoscenze sufficienti a capire se un edificio e un'infrastruttura possano resistere o no a una certa tipologia di scossa e abbiamo tutti gli strumenti per garantire la sicurezza sicurezza alle persone, anche in occasione di eventi sismici. Il Governo del cambiamento alla parola «prevenzione» deve sostituire per sempre la parola «emergenza».

Signor Presidente, onorevoli membri del Governo, colleghi, Mahle è un'azienda produttrice di componenti automobilistici con sede a Stoccarda, in Germania. La Mahle Componenti Motori Italia SpA è presente in Italia fin dal 1987, anno in cui ha acquisito il controllo della precedente società Mondial Piston SpA, attiva fin dal 1946. In Italia sono presenti due stabilimenti di produzione, uno a La Loggia (Torino) e uno a Saluzzo (Cuneo), per un totale di circa 500 dipendenti. Lo stabilimento di Saluzzo comprende il processo produttivo di fusione della lega d'alluminio, nonché prelavorazioni meccaniche di formatura del pistone, nel quale sono impiegati 200 operai e altri 40 lavoratori tra impiegati, quadri e dirigenti. Nello stabilimento di Saluzzo, nel 2018, il ricorso alla cassa integrazione ordinaria ha coinvolto un numero compreso tra i 50 ed i 200 operai sui 200 totali; come riferito dalle associazioni sindacali coinvolte, il piano industriale presentato dall'azienda tedesca non prevede adeguati investimenti in Italia, comportando un depotenziamento per i siti produttivi presenti sul territorio italiano. Nello stabilimento di Saluzzo, inoltre, vengono prodotti i componenti per motori diesel e tale settore risulta in contrazione, causando preoccupazione per il futuro dello stabilimento alla luce dei mancati investimenti su nuove produzioni. In generale, il mercato automobilistico europeo presenta forti contrazioni che rischiano di causare gravi conseguenze nel comparto industriale italiano e dell'Unione europea. In un incontro tra i rappresentanti sindacali della Mahle e i vertici della stessa, svolto il 7 dicembre 2018 presso l'assessorato al lavoro della Regione Piemonte, i dirigenti Mahle hanno illustrato la situazione economica nei vari stabilimenti europei dell'azienda, hanno ribadito la volontà di mantenere la presenza in Italia, ma non hanno fornito indicazioni sulla possibile diversificazione produttiva e sugli sviluppi futuri. Secondo quanto risulta all'interrogante, ci sarebbe il rischio di una completa riorganizzazione aziendale che comporterebbe una drastica riduzione produttiva negli stabilimenti italiani di La Loggia e di Saluzzo, con conseguente crisi occupazionale. Si chiede di sapere se il Ministro sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e se intenda convocare un tavolo presso il Ministero, affinché si possa avere chiarezza sui futuri piani industriali dell'azienda in questione, al fine di tutelare i livelli occupazionali attuali. sociali*. Signor Presidente, ringrazio il senatore interrogante. Riguardo alle problematiche evidenziate relativamente alla società Mahle, ricordo che l'azienda, con sedi in Germania a Stoccarda e in Italia a La Loggia (Torino) e a Saluzzo (Cuneo), è *leader* a livello mondiale nella produzione di componenti per motore e la sua clientela è costituita da gruppi automobilistici internazionali. In passato, l'azienda, aveva già fatto richiesta del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per lo stabilimento di La Loggia (Torino) e per una sede di Trento, con la contestuale stipula di un contratto di solidarietà, che ha stabilito per dodici mesi la riduzione massima dell'orario di lavoro settimanale, come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'industria metalmeccanica, per 182 lavoratori (su un organico complessivo di 799). Ad oggi, non risulta esservi alcuna richiesta di trattamento CIGS per la sede di Saluzzo (Cuneo), fermo restando - posto che l'azienda coinvolta opera specificamente in Piemonte - che la procedura potrebbe essere gestita anche a livello regionale. Tuttavia, alla luce di quanto esposto, dichiaro la totale disponibilità del Ministero dello sviluppo economico ad avviare un tavolo di confronto con le parti interessate, ovviamente con richiesta da parte dei soggetti coinvolti. Sotto il profilo degli interventi a sostegno delle imprese in Piemonte, colgo l'occasione per ricordare che il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Piemonte e Invitalia SpA hanno sottoscritto, a luglio scorso, un accordo di programma per sostenere programmi di investimento nelle aree di crisi industriale non complessa del Piemonte ed è in corso la conclusione dell'*iter* per il riconoscimento dell'area di crisi industriale complessa per il territorio di Torino, in cui è localizzata la maggior parte degli stabilimenti produttivi, per rilevanza e dimensione, della Regione, tra cui anche FCA.

quali riguarda l'attenzione che come maggioranza dobbiamo mantenere nei confronti di tutte le aziende straniere che controllano importanti *asset* produttivi italiani. È fondamentale che chi decide di fare investimenti nel nostro Paese garantisca l'adeguato impegno economico e la tutela dell'occupazione. Questo caso sottolinea inoltre la delicata situazione industriale nella Regione Piemonte, dove sono diversi i *dossier* di crisi aziendale aperti. Non a caso il Piemonte, secondo gli ultimi dati presentati dal MISE, è la quarta Regione italiana per domande di reddito di cittadinanza; si tratta, dunque, di una particolare e delicata situazione che merita la giusta attenzione da parte del Governo. Vorrei poi fare una mia osservazione personale per quanto riguarda il reddito di cittadinanza. Signor Ministro, se il reddito di cittadinanza funziona andiamo avanti su questa strada; siamo agli inizi e dobbiamo ancora vedere se è una misura che porta dei frutti, come spero e penso.

sia orgoglioso di quello che ha fatto, perché qualunque lavoro dà dignità, anche pulire i bagni.

Signor Presidente, Ministro, colleghi, premetto che l'Italia, per la sua tradizione industriale, possiede numerose storiche aziende che rappresentano l'eccellenza del *made in Italy* nel mondo e che tali aziende, grazie alla straordinaria qualità della loro produzione, sono riconosciute in tutto il mondo e il cosiddetto marchio associato, in molti casi, è divenuto patrimonio industriale mondiale. mondiale. Nel corso degli ultimi anni importanti marchi storici sono stati oggetto di operazioni di acquisizione da parte di multinazionali con sede e produzione all'estero all'estero e tali operazioni, in numerosi casi, hanno provocato il trasferimento della produzione all'estero, con conseguente chiusura degli stabilimenti storici, il licenziamento, nel corso degli anni, di decine di migliaia di lavoratori e la perdita di quel *know how* industriale che era frutto di un costante lavoro imprenditoriale e di ricerca tecnologica. Si consideri, inoltre, che, oltre ad un impoverimento del tessuto industriale, queste chiusure hanno provocato e provocano un impoverimento del tessuto sociale e culturale nelle zone su cui insistono tali stabilimenti e che le operazioni di acquisizione di importanti marchi storici italiani continuano anche in questi anni, come nel caso dell'azienda dolciaria Pernigotti di Novi Ligure (Alessandria), per affrontare la quale è stato peraltro attivato, presso il Ministero dello sviluppo economico, un apposito tavolo di monitoraggio per la salvaguardia dei livelli occupazionali. Alla luce di questi fenomeni industriali appare sempre più necessario un intervento a tutela dell'occupazione, dell'integrità dei marchi storici, della qualità della produzione e della salvaguardia del tessuto sociale, economico e culturale delle aree su cui insiste l'azienda. Si chiede pertanto quali misure il Ministro intenda adottare per la salvaguardia dei cosiddetti marchi storici italiani, prevedendo specifici strumenti normativi, e quali iniziative il Ministro intenda intraprendere per tutelare i livelli occupazionali dei lavoratori impiegati nelle storiche aziende italiane, oggetto di operazioni industriali che prevedono il trasferimento della produzione all'estero o in aree diverse dalle zone di origine dell'azienda.

per salvaguardare i livelli produttivi e la sopravvivenza stessa delle imprese italiane e per tutelare i lavoratori. Il decreto dignità, che ha il merito di aver dato un impulso positivo ai contratti di lavoro a tempo indeterminato, ha posto un freno alle delocalizzazioni delle imprese che abbiano ottenuto aiuti di Stato per effettuare investimenti. Abbiamo infatti introdotto l'obbligo di non trasferire per cinque anni in Stati fuori dall'Unione europea l'attività economica che ha beneficiato del sostegno pubblico, pena la decadenza dal beneficio e l'irrogazione di una specifica sanzione amministrativa. Lo stesso vale per imprese che vanno fuori dal territorio italiano, ma in quel caso c'è solo la decadenza dal beneficio, con interessi, e non l'irrogazione di una specifica sanzione. Con una misura contenuta nel decreto crescita, in discussione in Consiglio dei ministri tra poche ore, si introdurrà nell'ordinamento la definizione di marchio storico di interesse nazionale e sarà fatto un apposito logo per valorizzare le imprese titolari di questo marchio, sia per consentire la certificazione di azienda storica del *made in Italy*, sia per tutelarne i livelli occupazionali e la sua produzione. Il Ministero dello sviluppo economico avrà la possibilità di poter procedere d'ufficio all'iscrizione di un marchio nel registro speciale, nel caso in cui vi sia stata notizia che l'impresa intenda chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, qualora risulti che il titolare non abbia iscritto questo marchio nell'apposito elenco. Per salvaguardare i livelli occupazionali e per garantire la prosecuzione dell'attività produttiva sul territorio nazionale è stata anche prevista l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale (per accedere al quale occorrerà seguire un'apposita procedura). Per accedere al Fondo, previa iscrizione del marchio all'interno del registro, l'impresa dovrà notificare senza ritardo al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative ad un progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento, e dovrà individuare i potenziali acquirenti, informando periodicamente il Ministero dello sviluppo economico delle proposte di acquisto ricevute e fornendo una relazione per ciascuna di esse. potrà essere istituito un apposito logo dei «marchi storici di interesse nazionale», che le imprese iscritte nel registro potranno utilizzare per le finalità commerciali e promozionali. Questa è solo una delle iniziative di questo Governo per frenare le delocalizzazioni delle imprese italiane e tutelare i livelli occupazionali. In tale direzione, il mio impegno come Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali sarà sempre massimo, perché quando un'azienda delocalizza, porta fuori dall'Italia non solo gli impianti ed il proprio mercato, ma anche il proprio *know-how*, ossia quel bagaglio di esperienze e conoscenze accumulato negli anni con il concorso delle insostituibili maestranze italiane. *(Applausi Questa norma la dedichiamo ai lavoratori della Pernigotti, che sebbene non potranno godere dei vantaggi di questa norma perché non può essere retroattiva, l'hanno ispirata e non consentirà mai più altri casi Pernigotti.

Signor Ministro, siamo soddisfatti di questa risposta e ci rende felici apprendere che la salvaguardia del *made in Italy*, uno dei punti di forza

grazie a questo Governo che è al lavoro da meno di un anno e si sta impegnando in provvedimenti seri, per i quali non servono delle proposte di legge dagli *iter* veloci soltanto per

che casi come quello della Pernigotti e dei suoi lavoratori non si verifichino più.

e tanti altri ancora certificano che in Italia la crescita è negativa. Praticamente, siamo in recessione: il fatturato industriale è a -7,3 per cento, gli ordinativi a -5,3 per cento; aumenta la cassa integrazione e diminuisce la possibilità per le persone di avere un reddito pieno. A fine maggio, quando lei si è insediato al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero del lavoro (in sostanza quando siete andati al Governo), in Italia gli occupati erano 23.327.000; a febbraio 2019, gli occupati in Italia erano 23.211.000, cioè 116.000 lavoratori e lavoratrici in meno. Signor Ministro, la situazione è molto grave. È chiaro che la vostra ricetta non funziona. Ma c'è una situazione ancora più grave che è quella delle aree di crisi complessa. Sono 18 in Italia, distribuite su tutto il territorio, da Portovesme a Taranto, a Savona, a Trieste, a Gela, e così via dicendo, territori che hanno subito crisi devastanti nel corso dell'ultimo decennio: 60.000 lavoratori dislocati in queste 18 aree di crisi, da gennaio sono senza stipendio perché lei, il suo collega dell'economia, il suo Governo non avete avuto il tempo di fare un decreto. *(Applausi dal Gruppo PD)*. E non ci dica che ha firmato due giorni fa. Quello era un atto dovuto, ma il decreto non è ancora applicabile perché non porta la firma dell'Economia e la registrazione alla Corte dei conti. Allora, Ministro, sulla cassa integrazione state umiliando le persone; sulle aree di crisi avete una dote di 721 milioni di euro in gran parte della scorsa legislatura: perché non investite quelle risorse per dare continuità produttiva e creare lavoro? Dai territori ci arrivano forti lamentele forti ritardi nella realizzazione dei progetti di riconversione. Pensi che la Commissione industria del Senato ha avviato un'indagine sulle 18 aree di crisi: la settimana scorsa abbiamo completato l'area di Savona e la settimana prossima discuteremo per quella di Taranto. La domanda, Ministro, è semplice: a che punto è l'attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi complessa? Perché lei, ancora in questi giorni, non è in grado di dire come come si realizzano questi progetti e come effettivamente si costruiscono le condizioni perché le persone possano rientrare nel posto di lavoro, magari con progetti anche innovativi?

stime OCSE e quindi avremo modo di spiegare da tre punti di vista diversi i tipi di intervento che stiamo portando avanti. Prima di tutto ricordo che l'OCSE, a settembre 2018, ci chiedeva di non cancellare la cosiddetta legge Fornero. Adesso, in un nuovo *report* di questi giorni, scrive che bisogna abrogare quota 100, mostrando coerenza con ciò che ha sempre sostenuto ma non tenendo conto che quota 100 era un impegno preso sia dal MoVimento 5 Stelle che dalla Lega con gli italiani e noi abbiamo deciso di mantenere la parola data. credo sia sbagliato chiedere già di abrogare una misura che sta avendo grande successo e che avrà presto impatto sulla qualità della vita di tanti italiani. Inoltre, dal rapporto dell'OCSE emergono stime che evidentemente non possono considerare in modo adeguato le misure del Governo che si stanno mettendo in atto proprio in questi giorni, tra cui il decreto crescita e il decreto sblocca cantieri, che servono proprio a rispondere al momento di congiuntura economica difficile che sta attraversando l'Europa, che non era prevedibile e che risente degli scontri internazionali sul piano del commercio e dell'effetto della Brexit. Per rispondere puntualmente ai quesiti della senatrice interrogante parto dal fatto che presso il MISE ogni giorno parliamo con le imprese in crisi per garantire una rapida e positiva soluzione delle varie problematiche, la continuità produttiva e la salvaguardia dei lavoratori. Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, al Ministero di mia competenza abbiamo firmato il decreto con cui sono stati assegnati alle Regioni 117 milioni di euro per il 2019 per le aree di crisi complessa

Per quanto riguarda le ragioni dei ritardi nella realizzazione dei progetti per accedere al beneficio, ci sono vari aspetti: l'effettivo reperimento a cura dell'impresa delle risorse finanziarie complementari al contributo di legge, variazioni del programma e dell'assetto organizzativo delle imprese e la necessità delle imprese di realizzare i progetti in tempi più lunghi rispetto a quelli inizialmente preventivati, cioè alcune imprese stanno cambiando il cronoprogramma dei progetti che ci avevano presentato. In merito alle risorse stanziate per la copertura di tutti gli interventi programmati o in via di programmazione, tenuto conto dei progetti di conversione e riqualificazione industriale che riguardano aree di crisi industriale complessa, a questi interventi sono destinati complessivamente 283 milioni di euro. A queste risorse dovrà aggiungersi parte dello stanziamento previsto in legge di bilancio, per il biennio 2019-2020, per il finanziamento degli interventi ai sensi della legge n. 181 del 1989, destinati alla riconversione e alla riqualificazione produttiva delle aree industriali. Stiamo parlando di ulteriori 150 milioni di euro. Quanto alle istanze pervenute nel corso degli ultimi mesi, come richiesto nell'interrogazione, se per istanze si intendono le domande di agevolazioni trasmesse, si evidenzia che da dicembre sono pervenute 112 domande. Per quanto riguarda le richieste di avvio delle procedure di riconoscimento di aree industriali di crisi sono pervenute due istanze per il riconoscimento dell'area di crisi industriale complessa di Torino e di Massa-Carrara. Alla Commissione di competenza riconosco il lavoro meritorio sull'indagine conoscitiva che state portando avanti. Signor Presidente, la risposta del Ministro è superficiale, insufficiente e parziale. Emerge desolatamente quello che noi evidenziamo da mesi: la totale assenza di un'idea, una visione del sistema Paese. Ministro, in Italia la disoccupazione giovanile durante il vostro Governo è passata dal 32 al 32,8 I dati ci dicono che non avete abrogato la povertà, ma la dignità del lavoro sì. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Avete abrogato le politiche industriali, avete perso un anno prezioso,

questo è il sistema che crea lavoro. Invece di organizzare *tour* vacanza, Ministro, *(Applausi dal Gruppo PD)*dai *gilet* gialli, che predicano violenza e odio, vada nelle aree di crisi industriale complesse, vada a Taranto, dove l'aspettano dalle elezioni. dai lavoratori dell'Alcoa, non li costringa a venire sotto al Ministero per pietire il pagamento della cassa integrazione. PRESIDENTE. Concluda. e con quali risorse aggiuntive la reindustrializzazione. Ministro, lei festeggia il *memorandum* con la Cina; abbia a mente, durante questi festeggiamenti, che mentre lei cerca di raccattare qualche carretto per esportare arance nel terzo Paese produttore di arance nel mondo*,* la Francia vende 300 Airbus. *(Applausi dal Gruppo PD).* Ministro, un consiglio da una persona di una certa età. Noi vogliamo bene all'Italia. Ministro, studi e poi ci dica con quali politiche industriali voi volete affrontare i problemi del Paese.

ormai è tempo di un primo bilancio. Sono passati oltre dieci mesi dalla data in cui lei ha giurato come Vice*Premier*, Ministro dello sviluppo economico e Ministro del lavoro

ridotta, su pressione dell'Unione europea, all'1,1 per cento; siamo invece in piena recessione economica. Siamo in recessione economica da nove mesi si aggrava al punto tale che le ultime previsioni parlano per l'Italia, se va bene, di una crescita zero per quest'anno. Siamo l'unico Paese dell'Unione europea in recessione economica, con gli indici di caduta industriale a febbraio pari a

Tutti dati negativi che sono emersi anche in questo dibattito. Il collega della Lega ha parlato di un'industria importante di Saluzzo e lei ha risposto che aprirete un tavolo di crisi regionale. Sa quanti tavoli di crisi nazionali vi sono al suo Ministero? 153. Lei aveva promesso ai lavoratori della Pernigotti che avrebbe salvato l'azienda. Non le cito le dichiarazioni fatte dai lavoratori della Pernigotti, che sono irriferibili in quest'Aula. «Di Maio, tante promesse, ma ci ha snobbati scappando come un (...)» e le lascio immaginare. *(Commenti della a quella della Pernigotti, vi sono crisi industriali pesanti: da quella dell'Alitalia, per la quale avevate promesso una soluzione industriale e, invece, chiederete un nuovo rinvio, alla Piaggio, per cui lei dà soltanto la cassa integrazione ma non trova una soluzione industriale, a Termini Imerese, dove ormai è chiara quella che è stata una grande truffa, ma dove ancora lei non dà una soluzione industriale. Le chiedo perché le sue previsioni fossero clamorosamente sbagliate; perché l'11 gennaio di quest'anno è stato annunciato un miracolo economico e siamo, invece, in piena recessione economica, industriale e sociale, del lavoro dell'occupazione? Perché i vostri provvedimenti, secondo tutti gli osservatori, nazionali e internazionali, hanno effetti negativi sul tessuto industriale e sociale del Paese? finale, e mi collego con la Lega, è: quanto aspettate a cambiare politica economica in maniera drastica? Perché i cittadini italiani non hanno bisogno di diventare disoccupati per poter essere assistiti dai dai sussidi del reddito di cittadinanza. Hanno bisogno di un Ministero che sia davvero il Ministero dello sviluppo economico e non il Ministero della recessione economica.

che sul tema Pernigotti il Ministero è al lavoro con l'*advisor* proprio per trovare una soluzione per quei lavoratori e per fare in modo che questo non si verifichi più. Ma il problema della Pernigotti non è di delocalizzazione. Il problema è che vi è un soggetto straniero che ha comprato il marchio e lo stabilimento con i lavoratori. Ora, si vuole liberare dello stabilimento e dei lavoratori e tenersi il marchio. E noi invece vogliamo che quello stabilimento continui a produrre e che i marchi storici italiani non finiscano più nelle mani straniere proprio per questi comportamenti. Detto questo, la sua interrogazione, che riguarda prettamente le politiche industriali, mi permette di rispondere anche all'interrogativo finale della precedente senatrice interrogante che, invece, mi aveva posto domande sugli ammortizzatori sociali. Il tema vero è che lei dice, giustamente, che c'è un problema di crescita economica da nove mesi. Ma questo dimostra che è impossibile che, sin dal giorno in cui siamo entrati al Ministero, noi abbiamo causato un problema di crescita economica per questo Paese. *(Applausi dai Gruppi Se poi si vuole dare la colpa della crisi economica europea al Governo italiano, si faccia pure, tanto, c'è un lungo elenco di colpe che si attribuiscono a di tutto il mondo. Noi stiamo varando un decreto crescita proprio per affrontare questo momento di congiuntura economica difficile a livello europeo e internazionale, dovuto alla guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina e al tema della Brexit, che sta sfiduciando i mercati. Questo ha bloccato le esportazioni e, per questo, abbiamo firmato gli accordi con la Cina, che valgono fino a venti miliardi di euro per le nostre imprese che andando in quel mercato potranno esportare, sì, le arance, ma anche tanta altra eccellenza del *made in Italy* in un Paese ad alta domanda interna. precedentemente dei temi importantissimi, che io condivido, voglio dare qualche dettaglio del decreto crescita che stiamo per votare in Consiglio dei ministri, appena finirà il *question time.* Misure fiscali volte a favorire le imprese e i professionisti. Tra queste: il superammortamento, l'ulteriore deducibilità dell'IMU sui capannoni industriali, che va oltre il 60 per cento sui beni strumentali, interventi per la riduzione dell'Ires, il sisma *bonus*,

e L-SP-PSd'Az).* La misura per incrementare gli investimenti delle casse previdenziali nell'economia reale, un piano di grandi investimenti nelle ZES. Ci sono misure per il rilancio degli investimenti privati, come la riorganizzazione efficace del fondo di garanzia per le PMI per sostenere le misure di accesso al credito delle imprese, che hanno enormi difficoltà; la possibilità di intervento di questo fondo anche a garanzia di obbligazioni emesse dalle piccole e medie imprese (i cosiddetti minibond), le misure di sostegno e incentivazione alla capitalizzazione delle imprese, consistenti interventi a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare, misure per accelerare il completamento degli interventi previsti nei patti territoriali e nei contratti d'area. Ci sono le misure per la tutela del *made in Italy*, che sono quelle quelle che ho indicato prima sui marchi storici, ma c'è anche il programma da 140 milioni di euro per l'*export* del *made in Italy* nel mondo, che è la più alta cifra mai stanziata negli ultimi dieci anni per il sostegno al *made in Italy* sul mercato e ci sono misure nel settore energetico, che avranno un impatto sull'economia. Io credo che in questa fase in cui l'Europa - e *in primis* la produzione industriale della Germania - sta risentendo di questo momento di crisi, questo provvedimento, il decreto crescita, insieme al decreto sblocca cantieri, siano due provvedimenti che interpretano le preoccupazioni di quest'Assemblea e mettono mano a una serie di interventi per rilanciare l'economia

Ovviamente, interpretando quello che i telespettatori hanno ascoltato, non posso che dichiararmi profondamente insoddisfatto perché il Ministro non ha risposto alle domande. Ha fatto nuove promesse, ma non ha risposto alla domanda perché dopo dieci mesi siamo in profonda recessione economica, non come gli altri Paesi europei, perché nessun altro Paese tra i 28 Paesi dell'Unione è in recessione economica. Hanno tutti una crescita superiore all'1, 2, 3, 4 per cento nelle stime. *(Commenti dal Gruppo M5S).* Aggiungo di più, caro Ministro: l'Italia era già l'ultimo vagone nella crescita, questo ultimo vagone si allontana dagli altri, perché aumenta il divario con il resto dell'Unione europea. Lei, quindi, non risponde sui motivi per cui avete fallito e pretende di dare altre ricette per il futuro. Prima dica perché hanno fallito i suoi provvedimenti, perché non c'è stato affatto il miracolo economico, non c'è stato affatto l'aumento della produzione industriale, non c'è stato affatto l'aumento dell'occupazione. Ciò non è determinato soltanto dal fattore internazionale, che era prevedibile, perché ve l'avevamo detto che c'era una condizione internazionale negativa,

quindi, la recessione è dovuta a questi effetti, perché l'*export* lo scorso anno ha continuato a crescere, seppure meno rispetto agli anni precedenti. Si tratta quindi di un fattore interno che si somma ovviamente a difficoltà internazionali che non avevate previsto. Per quanto riguarda gli accordi sulla Cina, due miliardi - perché di due miliardi si parla negli accordi, a parte le aspettative - non sono nulla rispetto ai 30 miliardi firmati con un solo contratto dalla Francia che ha venduto gli Airbus e in Cina le nostre arance ci vanno da tempo, ci vanno via nave, perché andarci via aereo è del tutto improduttivo, perché costano troppo i voli aerei. Ministro, per favore, non siamo in campagna elettorale,

che anche la sinistra aveva cercato di attuare, lei li ripesca tentando di scambiarli per una nuova politica economica. L'unica politica economica di cui ha bisogno questo Paese è la riduzione delle tasse su chi lavora e su chi produce. L'unica politica economica di cui ha bisogno questo Paese è una politica industriale che lei non disegna nemmeno in quest'Aula perché non ce l'ha, perché il suo non è il Ministero dello sviluppo economico, è il Ministero della recessione economica, il suo non è il Ministero del lavoro, è il Ministero del sussidio. *(Commenti dal Gruppo M5S).* L'Italia ha bisogno di lavoro e produzione, non di sussidi

Signor Presidente, onorevole Ministro, i dati di tutti gli osservatori nazionali e internazionali indicano per l'Italia una situazione difficile, anzi, disastrosa: aumentano la disoccupazione e il debito pubblico con uno *spread* che ci rende costosissimo l'interesse sul debito pubblico; le aziende segnalano una flessione degli ordini; gli enti locali prevedono di aumentare le tasse e le tariffe a livello locale. Le previsioni che il Governo aveva rappresentato sulla nota di variazione al Documento di economia finanza nell'autunno sono completamente saltate. L'Italia è in decrescita, tutt'altro che felice. Vi preparate ad aumentare l'IVA fino al 25 per cento e le famiglie dovranno pagare. Il Governo sembra in uno stato confusionale: continuate ad attaccarvi l'uno con l'altro e a produrre norme di spesa disordinate; continuate a produrre debito che gli italiani dovranno pagare. Ogni giorno c'è una novità,

Nel contempo, però, il vostro impegno è concentrato sul creare disoccupati, con le chiusure domenicali, con la negazione dei *voucher*, con l'irrigidimento del Paese sempre più burocratizzato. Il vostro contratto prevedeva la *flat tax* con una revisione complessiva del sistema fiscale, che permettesse finalmente al Paese di liberare le capacità e la voglia di lavorare del popolo italiano. Fatto sporadicamente e in parte ha creato uno squilibrio nell'intero sistema. Onorevole Ministro, considerato l'attuale fallimento dei vari provvedimenti (dignità, concretezza e reddito di cittadinanza), cittadinanza), quale sarà l'azione che finalmente farà d'accompagnamento a una crescita del nostro Paese con un vero equilibrio fiscale e, quindi, il riordino complessivo con la *flat tax* (che era programma del centrodestra e, quindi, della Lega) e con una della famiglia seria con il quoziente familiare come annunciato solamente in conferenza stampa? Queste sono le azioni sulle quali chiediamo che il Governo investa. Glielo chiediamo dall'opposizione, prima da cittadini e poi da parlamentari.

sulle imprese in Italia sia fondamentale per favorire la crescita economica e il miglior modo per investire è abbassare le tasse. Ovviamente questi temi specifici sulla tassazione non sono

che in questo dibattito si citi spesso il fatto che la Francia abbia firmato degli accordi importanti con la Cina ed è per questo che ci siamo anticipati e li abbiamo firmati anche noi per evitare di farci battere, ancora una volta,

l'*export* e l'*automotive*. Questi due problemi si risolvono aumentando le relazioni commerciali verso l'Est del mondo per esportare di più e promuovendo l'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti sui dazi, in modo tale da permettere di nuovo le esportazioni di automobili europee verso quell'economia perché alcune volte, anche nelle automobili tedesche, quasi il 70 per cento è fatto di componenti italiani e, quindi, riguardano anche il nostro

medio significa aiutare le coppie giovani - ma anche quelle meno giovani - che fanno figli, agendo con un modello simile a quello francese, che inizieremo a introdurre gradualmente, che

Onorevole Ministro, lei è il Ministro dello sviluppo economico e, quindi, il sistema delle imprese e delle famiglie gravate dall'attuale organizzazione della tassazione è

Signor Presidente, sono contenta di fare quest'intervento oggi, visto che abbiamo parlato molto di *made in Italy*. «Il vino è uno dei comparti che può esportare molto nel mondo. È una delle nostre eccellenze e possiamo battere altri Paesi europei, anche nel mercato cinese»: così Luigi Di Maio alla vigilia del Vinitaly di Verona, nel confermare la sua presenza alla manifestazione del prossimo *weekend*. Ebbene, proprio di vino voglio parlare in questo mio intervento, per rendere edotti i colleghi di un'eccezionale occasione che il nostro Paese è chiamato a vivere in questo 2019. Mi riferisco al riconoscimento di «città europea del vino», che quest'anno è stato assegnato all'Italia e - precisamente - al Sannio, insignito del prestigioso riconoscimento dalla rete delle 800 città del vino presenti in 11 Paesi europei. La rete, formata dalle associazioni nazionali presenti negli 11 Paesi membri (Germania, Austria, Bulgaria, Slovenia, Spagna, Francia, Grecia, Ungheria, Italia, Portogallo e Serbia) copre un totale di quasi 800 città di tutta Europa. A partire dal 2012, inoltre, assegna annualmente il ruolo di capitale della cultura enologica del vecchio continente a un Paese dell'Unione, ponendolo al centro dell'attenzione e promuovendo in tale maniera l'attività culturale, l'identità, i paesaggi e i territori del luogo prescelto perché, come diceva il maestro Luigi Veronelli: «Il vino è il canto della terra verso il cielo». Il 2019 ha visto assegnare questo importante premio all'Italia e, tra le realtà che hanno proposto la propria candidatura, ha prevalso il territorio Sannio Falanghina, in particolare i Comuni di Castelvenere, Guardia Sanframondi, Sant'Agata dei Goti, Solopaca e Torrecuso, tutti della provincia di Benevento. Per me, quindi, è un reale piacere condividere con voi questo risultato che la mia terra ha conquistato meritatamente e mi preme ricordare che ad oggi il Sannio tutto, e non solo i Comuni che hanno fatto cartello sotto il nome Sannio Falanghina, è all'apice dell'Europa nel settore vinicolo, ottenendo riconoscimenti continui. Per questo mi auguro vivamente che in tanti decidano di visitare questi luoghi, di assaggiare i frutti della terra e, per quanto mi riguarda, mi fa piacere farmi portavoce di questo straordinario riconoscimento. Fatto dunque il mio invito, ci tengo anche a ricordare che lo scorso marzo la capitale europea del vino ha incontrato la capitale europea della cultura; infatti, a Matera, è stato presentato il progetto Biowine, che riguarda il trasferimento di buone pratiche per la tutela dell'ambiente in viticoltura e che coinvolge alcune importanti realtà del Veneto, della Campania e della Basilicata. Partendo da qui, dunque, il Comune di Matera ha proposto di impiantare filari di falanghina nei giardini del territorio per celebrare l'anno della doppia capitale europea e rafforzare il radicamento del binomio vino-cultura. Intanto, e chiudo, proprio al Vinitaly sarà presentato il programma dettagliato delle iniziative che si svilupperanno in tutto il 2019 per celebrare la capitale europea del vino che, con orgoglio, ribadisco essere il territorio della mia Benevento.